essere strategico per la nostra economia. Non si tratta solo di una questione economica: l'agricoltore e l'agricoltura sono soprattutto un grande valore da preservare; rappresentano da sempre le nostre tradizioni, la nostra storia e la nostra cultura; sono le radici di fatto del nostro Paese. Un valore così importante per la nostra filiera filiera alimentare, fattore fondamentale e indispensabile per tutte le eccellenze del *made in Italy*, ci rende orgogliosi e fa troneggiare il nostro Paese come *hub*, come punto di riferimento nel mondo. Ricordo a chi ci ascolta che l'Italia, il nostro grande e ineguagliabile Paese, ha un *record* mondiale di denominazioni di origine protetta (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP). Per questo il settore agricolo e agroalimentare rappresenta il comparto strategico fondamentale del passato, del presente, ma ancor più per il futuro dell'economia nazionale. E, forse più di ogni altro, presenta quel carattere di interconnessione capace di agire da moltiplicatore economico anche nel settore industriale, enogastronomico e soprattutto turistico; valore che, per fungere da volano strategico, necessita sempre più di politiche capaci di rafforzare l'*appeal*, ma soprattutto necessita di sostegno alla produttività, all'innovazione e al rispetto delle tradizioni, affrontando le sfide con la consapevolezza di essere il Paese *leader* sotto il profilo dell'agroalimentare. Questo è un approccio voluto dal Governo Meloni e portato avanti con passione e competenza dalla Commissione della quale faccio parte, la 9a Commissione, per la quale ringrazio il presidente De Carlo e il relatore Bergesio. comparto che - come è noto - sta attraversando un momento particolarmente complesso a causa della concomitanza di congiunture avverse, come il cambiamento climatico, il perdurare del conflitto in Ucraina, la diffusione di fitopatie. È una situazione di crisi che purtroppo determina gravi ripercussioni sul tessuto economico e sociale del nostro Paese, al quale il Governo Meloni ha inteso Alla luce di questa realtà il Gruppo che presiedo plaude al merito del ministro Lollobrigida e del Governo per aver dedicato quasi esclusivamente alle imprese agricole e della pesca l'intero provvedimento, un'attenzione che mai come in questa legislatura si è voluta porre al settore. un corposo provvedimento necessariamente all'altezza dell'importanza del settore, che prevede sostegno al lavoro in agricoltura, contrasto alle pratiche sleali e alla piaga del caporalato, stop alla diffusione della peste suina africana e alla brucellosi, nonché alla proliferazione delle specie alloctone come il granchio blu; ancora, misure per razionalizzare la spesa, migliorare l'efficienza del sistema informatico nel solco già tracciato da altre misure recentemente approvate, che hanno sancito la costituzionalizzazione dell'agricoltore custode del territorio, o permesso di incentivare l'imprenditoria giovanile agricola. Si tratta quindi di un provvedimento che nasce dal desiderio di ascoltare il grido di dolore delle imprese e delle associazioni del settore, pianificando interventi, investimenti e tutele, senza dimenticare la messa a terra delle ingenti risorse che il PNRR destina all'agricoltura. Dopo quattro lunghi anni, per esempio, si pone fine all'installazione selvaggia del fotovoltaico a terra, limitando ai soli terreni produttivi questo divieto; quindi, consumo di suolo zero per quanto riguarda il terreno fertile agricolo e nessuna speculazione. Sì, dunque, al fotovoltaico sulle coperture delle aziende agricole; no al fotovoltaico sul suolo agricolo, ciò al fine di di fermare anche le speculazioni dei grandi fondi di investimento che, in molte aree del Paese, stavano mettendo in difficoltà la produzione agricola, specie delle piccole e medie aziende agricole. sono poi il tema della fauna selvatica, che mi sta molto a cuore, e la battaglia per il contrasto alla peste suina, una piaga che necessitava di aiuti precisi ai nostri imprenditori, ai nostri allevatori, incentivando gli investimenti in termini di biosicurezza, andando a potenziare il fondo proprio dedicato con un rifinanziamento di cinque milioni di euro per il 2024 e di quindici milioni di euro per il 2025, permettendo anche l'utilizzo delle Forze armate e delle organizzazioni di volontariato e di protezione civile per contrastare il dilagante fenomeno della peste. Il tema che personalmente però mi sta più a cuore, signor Presidente, come a tutti noi e che ha colpito tutti gli italiani, è la lotta allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura: quella piaga odiosa, orribile e disumana che spesso si consuma nel silenzio, che è il silenzio di quei lavoratori, per lo più stranieri, pagati l'equivalente di un tozzo di pane che, nei campi di grano e pomodori, rischiano ogni giorno di perdere la vita per far fiorire le nostre eccellenze. Signor Presidente, vogliamo che l'orrore che tutti abbiamo provato per la morte di Satnam Singh non sia solamente un altro evanescente moto di indignazione generale popolare, ma diventi un esempio per dichiarare guerra senza confini allo sfruttamento in agricoltura. Stupisce il fatto che qualche organizzazione sindacale si renda conto solo ora del problema. Dov'era chi per anni avrebbe dovuto vigilare, tutelare e assistere i lavoratori del comparto? Signor Presidente, colleghi, noi non volteremo le spalle a chi quelle stesse spalle e mani le ha bruciate dal sole e dalla fatica per noi, per il nostro interesse. Con gli emendamenti a firma dei relatori, che come Gruppo abbiamo saldamente sostenuto, abbiamo posto le basi per la costituzione del sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, che coinvolgerà non solo i Ministeri competenti, ma anche tutta la filiera istituzionale, dall'Inps, che curerà anche la banca dati degli appalti in agricoltura, fino ad AGEA, potendo contare su una mole di dati che, incrociati tra loro, ci permetteranno di individuare già sulla carta le situazioni anomale e, quindi, poter intervenire con azioni mirate di prevenzione e contrasto. A noi piacciono i fatti e gli atti concreti. Per questo abbiamo chiare la visione e la strategia di contrasto al fenomeno, attuando concretamente efficaci forme di prevenzione. Solo così si sconfigge il caporalato, non di certo con la propaganda politica proprio di quella parte che, per anni - come ho detto - ha predicato bene e poi evidentemente razzolato male. Credo sia importante enunciare qui misure altrettanto efficaci come quelle relative al rafforzamento del ruolo del commissario per la siccità e al piano straordinario per riuscire a efficientare il sistema idrico italiano, nonché, come da riferimento alle imprese di interesse strategico nazionale, quelle per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva di Taranto, garantirne la sicurezza e disciplinare le procedure relative all'amministrazione straordinaria. La salute e il lavoro sono per il Governo Meloni una priorità non certo indifferibile. Il cuore del provvedimento riguarda dunque la nostra terra, la visione che vogliamo avere di un comparto fondamentale per la crescita del Paese, qual è quello agricolo. Sono questi i pilastri su cui far appoggiare le nostre certezze e quelle degli imprenditori agricoli, pur nella consapevolezza che la concorrenza dei prodotti esteri esteri è spietata, spesso anche sleale. Di fronte alle sfide di Paesi senza regole non possiamo e non dobbiamo arretrare di un millimetro, né ridurre la capacità produttiva dell'agricoltura europea e italiana. Al nostro comparto servono meno oneri fiscali inutili, meno burocrazia inutile e più controlli a carico degli agricoltori che sottraggono risorse al settore. Questa è la direzione e per questa ci stiamo battendo e ci batteremo, senza dimenticare il tema del libero scambio con i Paesi extra UE che producono prodotti alimentari e trasformano prodotti agricoli senza i vincoli che abbiamo qui in Italia.

alla nostra sicurezza alimentare. Signor Presidente, l'agricoltura è il DNA stesso del nostro Paese. Il Governo Meloni è dimostratamente sempre al fianco degli agricoltori e dei produttori; è dalla parte di chi lotta ogni giorno per difendere il *made in Italy* e l'agricoltura italiana. Noi questo lo condividiamo profondamente come Gruppo.

Signor Presidente, il provvedimento che stiamo per votare contiene norme importanti in materia di finanziamenti, di tutela del lavoro e di minore burocrazia e prevede una serie di interventi volti a fronteggiare situazioni di crisi. è quindi, sotto molti aspetti, un provvedimento condivisibile e di aiuto per l'agricoltura, primo custode dell'ambiente. Di questo impegno va giustamente e correttamente dato atto al ministro Lollobrigida e al Governo. In questa cornice, come Gruppo Per le Autonomie, avevamo presentato in Commissione una serie di emendamenti legati ad alcune specifiche problematiche del territorio che rappresentiamo. Purtroppo nessuno di questi emendamenti è stato accolto. Eppure, si trattava di proposte che, con un minimo di attenzione in più, potevano tranquillamente essere inserite nel testo, senza stravolgerne l'impatto o richiedere particolari ulteriori impegni di spesa. Mi riferisco in particolare al rifinanziamento del fondo per il bostrico: la disposizione, così come approvata, sembra voler escludere le Province autonome, che originariamente erano incluse e che sono quelle maggiormente colpite dal fenomeno; fino alle norme sui guardacaccia, che sono anch'essi pubblici ufficiali a tutti gli effetti e vigilano sulla tutela del territorio. Parlo di problemi che possono apparire marginali rispetto ad alcuni grandi temi, ma che impattano in maniera significante sull'agricoltura delle nostre Province. Penso si sia persa un'opportunità per licenziare un provvedimento più completo e all'altezza delle numerose sfide ed emergenze che la nostra agricoltura, in tutte le sue articolazioni, è chiamata ad affrontare. Come sa, Presidente, nel nostro Gruppo convivono differenti provenienze politiche e, quindi, ciascuno si esprimerà a modo proprio sulla questione di fiducia. Di certo, pur riconoscendo la bontà di molte norme, non possiamo non notare le criticità, a partire dalla mancata attenzione rispetto ai temi e alle problematiche di cui il nostro Gruppo si è fatto carico, che tuttavia ci auguriamo possano essere risolti nei prossimi provvedimenti, anche attuativi.

voglio ringraziare senza fingimenti il sottosegretario La Pietra e i relatori Bergesio e De Carlo per l'attenzione che hanno prestato alle richieste delle opposizioni. Ieri ho letto un'importante comunicato del ministro Lollobrigida, secondo cui con questo provvedimento si delinea quella che lui definisce l'agricoltura della Nazione. A me preoccupa che questa sia l'agricoltura della Nazione. Lo dico perché quello in esame è un provvedimento che non guarda al futuro, futuro, ma lascia completamente inalterate tutte le grandi sfide tecnologiche che la futura agricoltura dovrà C'è un progetto Fastweb con alcuni produttori di frutta del senese, che con i droni individuano e monitorano gli alberi e valutano l'impiego di eventuali fitofarmaci e quando irrigare le piante. Di tutto questo, del futuro, del bisogno di tecnologia, del bisogno di investimenti per gli agricoltori in questo provvedimento non c'è Non c'è neanche il superamento di alcune emergenze. Non sono state valutate tutte le criticità relative ai patogeni che stanno fortemente mettendo in ginocchio la nostra agricoltura e che dovrebbero stimolare l'avvio di una riflessione più completa sui cambiamenti climatici, al fine di emanare un provvedimento, insieme al Ministero dell'ambiente, che guardi Grazie, finge di guardare al passato, sapendo che più di tanto non si può fare, perché per fortuna la modernità è andata avanti nonostante gli intendimenti di questo Governo. Parto da tre punti. punti. Durante la campagna elettorale per le europee, un importante sindacato di agricoltori si è presentato, con le sue belle divise gialle, ai confini del Brennero dicendo che là non passerà più nessun prodotto e, accusando un'altra importante associazione di agricoltori, insieme ai grandi trasformatori e ai grandi produttori alimentari del nostro Paese, di essere responsabili di fare accordi per quella che loro definiscono agricoltura sleale.

Invece il silenzio è stato rotto dalla norma contro le contraffazioni contenuta in questo decreto, che oggettivamente sposa quella linea. Ciò mi ha stupito molto. Diciamo in maniera trionfale

Il secondo punto che a me ha molto stupito: c'è una mancanza di visione. Ripeto: a parte delle piccole sovvenzioni in in piccoli settori, non c'è una visione d'insieme di come portare l'agricoltura nel futuro tecnologico, come dicevo prima. Ci sono sempre più emergenze ambientali

è avvenuto. Visto che non c'è stata attenzione verso l'impresa agricola, mi aspettavo che ci fosse almeno attenzione rispetto agli imprenditori che in questo momento stanno attendendo le autorizzazioni per le rinnovabili. Possiamo pensare che le rinnovabili non siano il futuro - non sono così innamorata del *green* da non vederne i limiti - ma percepisco anche che siamo arrivati a una crisi energetica senza avere un adeguato e maturo *mix* energetico. Visto che abbiamo ottenuto 90 milioni per avere dei progetti

quell'articolo perché si parlava di terreni agricoli. Quindi, avete sottolineato che si possono fare le rinnovabili, in particolare il solare a terra, nelle cave e nelle discariche.

se richiedo un terreno per fare il solare, devo avere da subito la locazione (sei più sei). Voi sapete che prima si chiede il terreno e, nelle more dell'autorizzazione, quel terreno viene più o meno impiegato; non è detto che venga dato: se non c'è l'autorizzazione, quel terreno verrà utilizzato per altro. Aver subito previsto la firma della locazione comporta che un proprietario si troverà di fronte a un bivio: darlo a chi vuole produrre energia, con il dubbio che poi questo avvenga, o continuare nella produzione. Nel dubbio, voi sperate nella seconda scelta e non nella prima. Ancora una volta c'è un divieto velato velato verso un mondo che ha fatto degli investimenti. Fino a ieri si era detto che quello era il futuro ed era il modo con il quale si sarebbe superata la futura crisi energetica, perché di crisi energetiche, ahimè, ce ne saranno di continuo. Allora mi è venuto da sorridere nel leggere il comunicato del ministro Lollobrigida, perché ho pensato che, quando vi siete insediati due anni fa, nello *storytelling* per chiedere la fiducia a questo Parlamento avete iniziato dicendo che è finita la politica dei no,

delle promesse mirabolanti sul ritorno al nucleare o su un grande ponte, che però poi non è sovvenzionato e supportato in maniera pratica, poi alla fine nei vostri provvedimenti ci sono continuamente dei no, dei no, che vanno verso la produzione industriale e verso un modo nuovo di intendere questo Paese, forse, banalmente, più moderno. E, allora, anche se non aveste messo la fiducia, io avrei chiesto al mio Gruppo di votare contro questo decreto-legge perché non è il provvedimento che mi aspettavo per un comparto così importante come quello agricolo. I

istantanee e in due anni è stato fatto veramente il delirio, nel senso del nulla, salvo poi sentire lo stesso commissario dire che a Tortona e a Roma non ci sono più cinghiali. Vorrei che facesse una passeggiata a Roma,

e che in grandissima parte non offre la possibilità di una discussione in cui si cerca di capire. Vorrei partire da un dato. Ieri sono stato qui - eravamo in pochi,

in merito alla decretazione è una questione democratica, per quanto ci riguarda, che inerisce al ruolo partecipativo: utilizzare continuamente la decretazione e la fiducia mortifica il Parlamento e quindi

visto e considerato che da anni si va avanti in una situazione di grande difficoltà, in una grande impresa come Ilva. Siamo però al settimo decreto e, se non c'è alcuna prospettiva,

non solo non si tengono aperti gli impianti, ma non si può pagare e dare risposta all'indotto, a meno che l'indotto non lo facciamo saltare

penso che il Governo, cioè in questo caso il pubblico, debba prendere in mano la situazione e dire come intende andare in questa direzione, e in tal caso, coinvolgere i privati in una discussione per partecipano o no a un indirizzo, ma ci vuole un'idea del pubblico prima. Non si può andare continuamente alla cieca. Su questo non

Oggi la nostra agricoltura regge in quanto migliaia di lavoratori prendono 3, 4, 5 euro l'ora e magari in nero.

su come interveniamo e quindi modifichiamo questo stato di cose, perché ho cercato di dimostrare con i numeri quante sono le aree in tutto il nostro Paese. Ad esempio, si dice che il caporalato è

e, se salta questa realtà, salta un modello, che è fatto su questa impostazione. C'è un modello sistemico che va affrontato.

si oppongono al decreto-legge in esame, come si oppongono a tanti provvedimenti. Certo, nessuno pensava che questo testo potesse dare risposte addirittura definitive a problemi annosi e a tutti i problemi che riguardano l'agricoltura. in esame è il classico esempio di provvedimento necessario, che fa fronte a temi che richiedono risposte urgenti, per dare soluzione a disposizioni già vigenti, quindi continuare in una normativa positiva che possa dare le risposte che ci vengono chieste dal mondo agricolo. Per questa ragione esso contiene sia norme in materia di agricoltura sia norme che affrontano l'annosa questione dello stabilimento Ilva, che certamente non ha inventato questo Governo. Allo stesso modo, purtroppo, la morte del giovane lavoratore agricolo indiano Satnam Singh, che ha colpito e ha lasciato tutti noi in uno sconcerto terribile, pensando che una cosa del genere non potesse accadere, ha però messo in evidenza, purtroppo, nella sua triste e disumana brutalità, il problema del caporalato. ulteriormente e opportunamente intervenuto in Commissione sul tema dello sfruttamento dei lavoratori invisibili, che non sono solo stranieri. Non che questo faccia la differenza, ma ci deve far riflettere. ma ci deve far riflettere. Tuttavia, le norme per contrastare quella che è a tutti gli effetti una concorrenza sleale tra aziende agricole sane e aziende che non lo sono, o che comunque non rispettano la normativa, Nel corso dell'esame in 9a Commissione sono state approvate nuove disposizioni che mirano a contrastare il caporalato, aumentando i controlli di prevenzione e lo sfruttamento lavorativo, così come il lavoro sommerso e irregolare, sviluppando un'apposita strategia di contrasto. Certo come ci ha detto anche ieri il Ministro - si tratta di un inizio, non è una risposta definitiva e non è certo la soluzione al problema in modo definitivo. Ci sono norme che puntano anche a rafforzare i controlli in materia di lavoro e di legislazione sociale nel settore agricolo. E sono state approvate disposizioni per gli ammortizzatori sociali in agricoltura volti ad affrontare le emergenze stagionali. Il decreto-legge era nato dall'esigenza di prevedere interventi per sostenere il lavoro e contrastare pratiche sleali in agricoltura. da parte della Commissione ha aggiunto anche un articolo che prevede il rafforzamento delle sanzioni nel settore alimentare, ma il provvedimento è stato anche l'occasione per affrontare altre tematiche assolutamente urgenti: fermare la diffusione della peste suina africana e la brucellosi, limitare la diffusione e la riproduzione del granchio blu, ottimizzare la spesa, migliorare l'efficienza del sistema informatico agricolo nazionale e rinforzare i controlli nei settori agroalimentari e faunistico-venatori. Per le altre imprese agricole sono previste misure per affrontare le emergenze climatiche, contrastare la scarsità d'acqua e potenziare le infrastrutture idriche, posto che le aziende - lo sappiamo tutti - sono ormai il motore dell'economia agricola. Viene prevista la sospensione della rata dei mutui per la parte capitale, come accade in tante altre situazioni, o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura quando si verifica una drastica riduzione di fatturato. Viene altresì rimodulato, secondo le esigenze, il credito d'imposta riconosciuto per il 2024 a favore delle imprese attive nel settore della produzione di prodotti agricoli, della pesca o dell'acquacoltura che acquistano beni strumentali destinati a strutture produttive della ZES. Considerati i danni causati dalle alluvioni del 2023 in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, viene ampliata la platea dei datori di lavoro agricoli nelle zone colpite cui spettano le agevolazioni contributive. Anche questo è un importante risultato. Un nostro emendamento consente poi un più puntuale riconoscimento dei danni per le mancate produzioni causate dalle alluvioni lo scorso anno, utilizzando i fondi della gestione commissariale. Viene affrontata dal decreto-legge e dalle modifiche parlamentari la questione dell'installazione di pannelli fotovoltaici con disposizioni puntuali in zona agricola, ma anche con deroghe per l'attuazione del PNRR in determinate zone demaniali o pubbliche. A proposito di Piano nazionale di ripresa e resilienza, abbiamo avuto la notizia che l'Italia ha già ottenuto il via libera della Commissione europea per la quinta rata di 11 miliardi. L'Italia ha intanto già richiesto la sesta rata ed è stata gratificata con una rata maggiore proprio perché ha persino anticipato alcuni *target* previsti dalla settima rata per gli interventi nella lotta all'evasione fiscale. In tema In tema di pannelli fotovoltaici, i nostri emendamenti chiariscono il concetto di impianti fotovoltaici con moduli a terra estesi su aree agricole in modo ragionevole. È evidente che il modo ragionevole va sempre calato nella realtà. poi tutta la parte che riguarda le aziende in crisi, in particolare l'Ilva, come già ricordavo, con misure per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell'acciaio. Credo che siamo tutti concordi sia un tema che deve stare a cuore a tutti e che questa produzione e questa presenza devono assolutamente continuare. In conclusione, si tratta di un complesso di norme e di modifiche al decreto iniziale che auspicavamo

della Costituzione. La risposta è stata che si tratta di un decreto d'urgenza. In questa legislatura si procede per decretazioni d'urgenza. È una presa in giro intollerabile, che tutti stiamo notando. Il Quirinale vi sta ripetutamente mettendo in guardia ma voi state facendo un braccio di ferro. Inserire nel titolo degli articoli e dei capi la parola «urgente» non è altro che una distorsione della realtà per mettere in campo quello che è un vero e proprio abuso di potere, una prova di forza che lede alla base il principio della democrazia. Vediamo quali sono le urgenze. Di davvero urgente è forse solo quanto contenuto nell'articolo 1, cioè la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui per le imprese che hanno subìto una riduzione del volume di affari di almeno il 20 provvedimento è stato chiesto giustamente a gran voce da tutti. Noi abbiamo anche riportato l'*alert*, presentato in Commissione dall'ABI (Associazione bancaria italiana), circa la trappola insita nel provvedimento e cioè che le aziende che accedono a questa sospensione del mutuo possono incorrere in problematiche legate alla definizione della loro posizione debitoria, cioè potrebbero essere inserite tra le aziende deteriorate: aspetto molto importante sul quale abbiamo depositato un ordine del giorno che però non è stato accolto. Andiamo avanti tra i commi e gli articoli del decreto-legge. Appare chiaro che la gestione ordinaria, ponderata e condivisa non possa esistere per questo Governo. Infatti, si gestiscono si gestiscono le problematiche lasciando le patate bollenti ai commissari straordinari, che in questo decreto-legge sono ben due: uno per la zoonosi della brucellosi e l'altro per la diffusione spropositata del granchio blu. Poi c'è da capire perché per il secondo, il commissario per il contenimento del granchio blu, siano stati stanziati 10 milioni e per il primo nulla. La risposta fornitami non mi è stata chiara, ma c'è da dire che noi, come MoVimento 5 Stelle, già nel decreto *asset* abbiamo insistito per un piano di contenimento del granchio blu e adesso vedo che dopo un anno vi siete decisi a proporlo. Ancora, si procede con le disposizioni urgenti e questa volta per il sostegno del lavoro in agricoltura. È un altro grande tema che non può non essere affrontato con il mezzo della decretazione d'urgenza. L'urgenza si potrebbe ravvedere nelle azioni da mettere in campo per dare dignità ai lavoratori sfruttati per le interminabili ore sui campi di raccolta infuocati; parlo delle criticità legate al caporalato e alla sicurezza sui campi agricoli per lavoratori troppo spesso lasciati senza nessuna tutela Invece, proprio questo aspetto il Governo l'ha inizialmente dimenticato ed è dovuto ricorrere agli emendamenti del relatore una volta che le terribili notizie di cronaca hanno imposto di attenzionare quello che colpevolmente si stava tralasciando. Così è apparso un emendamento che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato: uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e regionali. Alla sua costituzione è scritto che concorrono il Ministero del lavoro, il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'Inail, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Agea e l'Istat, finalmente dialogano tra loro, ma è un provvedimento che noi parlamentari - come tutti voi fuori da questi palazzi - recepiamo facendoci solo un'idea di cosa sia. Ha tutta l'aria di un annuncio vuoto, buttato nel decreto in tutta fretta, non prevedendo nessun impegno di spesa o programma, affinché possa essere davvero operativo. modo vi è la banca dati degli appalti in agricoltura, a cui si iscrivono le imprese che intendano partecipare ad appalti richiesti dalle imprese agricole: sicuramente un mezzo utile alle imprese sane, in un mondo ideale, ma non di certo un modo per far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento. Anche questo credo sia stato buttato lì senza alcuna forza operativa. Dobbiamo augurarci che con il tempo il tutto possa prendere forma, ma intanto la soluzione urgente non l'abbiamo trovata. Altro articolo urgente è il 3, che è quello dei ristori, che dovrebbe correre in soccorso degli agricoltori in ginocchio a causa delle varie fitopatie, quale la moria del kiwi, la peronospora o la flavescenza dorata; peccato che, ad esempio, per la peronospora, in urgenza l'anno scorso, abbia stanziato solo un milione, poi aumentato a sette milioni: il nulla. L'urgenza, quella vera, è passata così. Gli agricoltori che hanno subìto i danni da queste fitopatie hanno dovuto risollevarsi da sé. Penso ai viticoltori che hanno visto marcire le piante prima della scorsa vendemmia ed in questa vendemmia forse nemmeno ci sono arrivati, visti i danni ai tralci. Stanziare delle cifre *spot*, tra l'altro in alcuni casi dagli importi assolutamente risibili, quali anche i quattro milioni per la moria del kiwi, è un comportamento da spot elettorale decisamente fuori luogo. Sulla questione della moria del kiwi, la scorsa legislatura, ad esempio, si è fatto un lavoro di approfondimento con un affare assegnato, poi conclusosi con una risoluzione che potrebbe ancora oggi essere d'ispirazione per l'attuale Governo. Non si possono inseguire le emergenze. Servono indagini approfondite con linee di ricerca specifiche, partendo da una mappatura della diffusione delle fitopatie supportata da un costante monitoraggio e valutazione degli effetti delle nuove pratiche agronomiche messe in atto e soluzioni varie per la definizione di linee guida di coltivazione, a cui dare poi la più ampia divulgazione. All'articolo 4 si passa al contrasto delle pratiche sleali. Si punta alla determinazione del costo medio di produzione da parte di Ismea, dato che da sempre presenta enormi criticità e che nei fatti non ha mai contenuto la spropositata forbice che c'è tra il prodotto tra il prodotto venduto sul campo e quelli sugli scaffali dei supermercati. L'ortofrutta subisce un ricarico di circa il 300 per cento rispetto alla cifra corrisposta ai produttori. Per non parlare degli squilibri che si registrano nel settore cerealicolo, versante trainante delle produzioni del *made in Italy*. Queste evidenze, insieme alle recenti proteste del mondo agricolo di tutta Europa, mostrano inequivocabilmente che i tempi sono maturi per specificare in maniera chiara cosa si intende per costo di produzione. È necessario specificare che nel costo di produzione entrano in gioco delle componenti che non possono essere trascurate, quali la collocazione geografica delle colture, le caratteristiche territoriali, le tecniche di produzione medio-ordinarie, il differente costo della manodopera negli areali produttivi. Parlando dei campi di grano, vengono subito in mente i cospicui danni generati dai cinghiali, situazione ora aggravata dalla diffusione della peste suina africana. Nessuno ha le bende davanti agli occhi, ma la militarizzazione degli interventi non è una risposta strategica. Serve professionalità nel rispetto dell'ambiente e nel contenimento degli elementi di contaminazione, altrimenti rischiamo danni peggiori, con la trasmissione della malattia alla filiera suinicola. Inoltre vergognoso è stato il tentativo di inserire emendamenti sulla caccia per tener fede ad accordi politici bellamente rivendicati dal deputato Bruzzone, fiero di definirsi grande cacciatore e dunque portatore di interessi personali e di settore, completamente fuori luogo nel decreto agricoltura. Riguardo alla caccia al cinghiale effettuata entro la mezzanotte con i visori notturni c'è la nostra ferma contrarietà, perché rappresenta un accanimento solo ai fini del godimento di quello che non è uno sport, ma un macabro gioco ad alta pericolosità per tutti. Meno male che riguardo all'istituzione del dipartimento per le politiche del mare non si parla di urgenze, visto che parte proprio in ritardo. Va a sostituire una struttura di missione già esistente in seno alla Presidenza del Consiglio, con la scusa che entro il 31 luglio bisognerà provvedere all'aggiornamento del piano del mare. Realisticamente entro tale data non si riuscirà nemmeno ad avviarne le strutture organizzative, ancor più vero considerati i tempi biblici di altre esperienze di gestione e realizzazione di questo Governo. Insomma, sembra l'ennesima norma *ad hoc* per rimpinguare la corte dei miracoli al servizio dell'Esecutivo. Un punto a favore va dato riguardo all'istituzione del Granaio Italia, cioè l'attivazione del registro telematico che permetterà di avere dati certi riguardo all'acquisizione e alla vendita delle produzioni cerealicole da parte di tutti i soggetti della filiera. Esso rappresenta anche uno strumento indispensabile per monitorare le giacenze dei cereali e dunque per riportare trasparenza sui mercati e tutelare le produzioni *made in Italy*. È una proposta che risale alla scorsa legislatura, sostenuta dall'ex deputato del MoVimento 5 Stelle Cillis con un suo emendamento di modifica alla legge n. 178 del 2020 in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole. Riguardo alle misure sulla scarsità idrica - vado a concludere - ci sarebbe tanto da dire, ma conteniamo giustamente i tempi. Viene da interpretare l'articolo sulle misure per la scarsità idrica come un sollecito che il Governo fa a se stesso e agli organismi che ha creato rispetto alla necessità di individuare le misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica. Peccato che queste erano tutte attività che dovevano essere espletate sin dall'emanazione del decreto legge siccità, che risale a 14 aprile dell'anno scorso. Dunque già entro metà maggio dell'anno scorso la cabina di regia avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve tempo alla crisi idrica. Secondo l'ultima relazione annuale dell'ARERA, nel nostro Paese il 23 per cento delle acque reflue è potenzialmente destinabile al riuso, ma ne viene effettivamente riutilizzato solo il 4 per cento in agricoltura. Questi sono i dati che devono far accendere le lampadine sugli impegni di spesa, e invece qui si va in urgenza a finanziare provvedimenti *spot* per far passare il messaggio che si lavora al problema della siccità ora con 15 milioni per la Sicilia, dove mancano proprio le infrastrutture. Non serve un giocoliere dei milioni; il ministro Lollobrigida li sposta con disinvoltura, così come i 30 milioni per la xylella sottratti ai distretti del cibo. Ma sicuro che il gioco vale… Grazie, Presidente, Presidente. Questo giocare a spostare i milioni vale la candela o non sfuggirà di mano al Governo? Accontentare con la fuffa non porta alla lunga i risultati, ma porta allo scasso. *(Applausi)*.

Il decreto-legge oggi in approvazione mette in campo circa 600 milioni di euro di risorse supplementari per i prossimi tre anni, 150 milioni per l'ex Ilva e il resto per l'agricoltura, con una lunga serie di interventi ampi e diversificati che spaziano dal credito d'imposta per gli investimenti sulle ZES agli incentivi per la copertura totale o parziale degli interessi passivi pagati dalle imprese agricole e per accedere ai finanziamenti bancari. Una tutela importante su questo tema, signor Presidente, perché sappiamo quante aziende agricole sono in difficoltà come sappiamo della mancanza di produzione e di redditività. Questo provvedimento è una buona notizia per il settore primario, segno dell'attenzione del Governo, del Parlamento e della Commissione di cui facciamo parte verso gli agricoltori quali custodi dell'ambiente e del territorio, depositari di tradizioni millenarie. Molteplici gli obiettivi, che vanno dal sostegno alle imprese in difficoltà agli indennizzi per le emergenze, dalla trasparenza nei mercati all'utilizzo consapevole del suolo agricolo, dal contrasto alla peste suina africana (PSA) al contenimento del granchio blu e al contrasto alla brucellosi e tubercolosi, senza tralasciare gli interventi a tutela dei territori colpiti dalla siccità e soprattutto del sistema assicurativo, che va naturalmente rivisto. Vi è poi l'introduzione di misure per un più efficace contrasto al fenomeno del caporalato, a partire dall'istituzione di un sistema informativo pubblico dove saranno condivise le informazioni degli organismi statali e regionali, a partire da INPS, Inail, Ispettorato nazionale del lavoro, collegandosi con Agea con un *database* informatico organico per prevenire e combattere gli abusi. La piaga del caporalato va debellata; sicuramente non vi si riesce solo con questi emendamenti al decreto, però sono un primo passo importante, per cui riteniamo, come relatori, di aver fatto il nostro dovere inserendoli nel provvedimento. *(Applausi)*. È stato poi approvato un emendamento, che ritengo di fondamentale importanza, sull'operatività di Granaio Italia, che permette la registrazione informatizzata delle operazioni di carico e scarico dei cereali: una misura volta a garantire la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare. I nostri produttori e gli agricoltori sono vessati dalla concorrenza di prodotti che arrivano dall'estero. Non c'è trasparenza, non c'è chiarezza e con questo sistema riusciamo a monitorare meglio la situazione. Abbiamo lavorato poi tutti insieme ad alcuni correttivi della disposizione relativa alla limitazione all'uso del suolo agricolo, per un suo uso consapevole, soprattutto con il divieto di installare gli impianti fotovoltaici con moduli collegati a terra nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici.

ai moduli sollevati, ma neppure agli impianti a terra in cave, miniere, in aree in concessione a Ferrovie dello Stato e aeroporti. Insomma, si è tutelata ancora una parte del decreto

Rientra sempre tra le azioni volte alla trasparenza, alla tracciabilità del mercato, al contrasto alle truffe e alle false denominazioni, l'emendamento a prima firma del vice presidente Centinaio e di tutta la Lega che rende tracciabile il vino, dalla vite alla bottiglia, con il collegamento tra lo schedario viticolo e i registri dei produttori vitivinicoli. Tale misura è volta a far sì che in questo settore, così importante per il nostro Paese,

a favore degli allevatori di specie di razze autoctone iscritte al libro genealogico e a rischio di estinzione. Parliamo della razza piemontese, della chianina, della romagnola, della maremmana, della marchigiana e della podolica, più alcune pochissime razze a rischio di estinzione. È un passaggio fondamentale, molto atteso dai 10.000 allevatori di questo settore che sono in gravissima difficoltà. Il tema delle vacche nutrici che ogni anno diminuiscono è sintomo di non avere più garanzia per il futuro di quell'8 per cento di consumo di carne bovina italiana prodotta da razze italiane che abbiamo fino ad oggi.

Governo per arrivare anche qui ad una tracciabilità certificata certa e importante. A questo è stato collegato il fondo di sviluppo delle filiere, con ben 32 milioni di euro di stanziamento destinati ai produttori di grano duro per finanziare i contratti di filiera

contro la diffusione del granchio blu che è veramente un dramma per i nostri pescatori e rappresenta un tema che va affrontato con decisione. La nomina del commissario sicuramente contribuirà su questo fronte. il contrasto alla peste suina africana, come abbiamo detto più volte, dobbiamo proteggere il settore suinicolo nazionale, che va dall'allevamento ai prosciutti, ai salumi, ai culatelli e a tutti quelli che sono i prodotti straordinari della salumeria italiana, che vale 20 miliardi. Si rende necessario a tal fine un intervento strutturale. Lo dico a lei, Presidente, e, per suo tramite, voglio trasmettere alla senatrice Naturale che ha parlato poc'anzi, noi non siamo assolutamente d'accordo sul fatto che il nostro collega Bruzzone agisca per interessi personali perché questo non è assolutamente vero. *(Applausi)*. Io le chiedo anche di chiedere scusa perché sappiamo tutti bene che la legge n. 157 del 1992 è ormai superata. Parlavamo di milioni di cacciatori mentre oggi sono poche centinaia di migliaia. Coloro che possono intervenire direttamente sono meno di 100.000 per dare una mano a questo settore. Allora con l'utilizzo consapevole di un contingente specializzato di 177 unità del personale delle Forze armate per l'attuazione dei piani di controllo e soprattutto per dare una mano al settore e limitare i danni della PSA perché l'eradicazione è complicata e difficile e dobbiamo arrivarci in questo modo,

Qui avremo la possibilità di abbattere e di catturare questi benedetti capi infetti che stanno contagiando in modo drammatico molte Regioni, tra cui quella da cui provengo, che è la Regione Piemonte, dove si trova anche un patrimonio suinicolo molto importante.

immagini dell'alluvione che in questi giorni ha colpito il Piemonte e la Valle d'Aosta. In appena sei mesi l'Italia è stata devastata da oltre mille eventi estremi tra laghi e fiumi in piena al Nord, siccità al Sud, 257 grandinate anomale dall'inizio dell'anno, 86 86 trombe d'aria, 10 valanghe, 25 fulmini con vittime e danni e 611 nubifragi. Questi sono dati dell'Osservatorio europeo, non sono dati stimati da qualche giornalista. una priorità quella di individuare le strategie per ridurre i danni e tutelare le colture. L'ha detto bene ieri anche il ministro Lollobrigida e lo condividiamo, perché perché purtroppo - lei lo sa bene, Presidente - che il ristoro dei danni in agricoltura ad oggi è ancora molto variabile e non quantificabile. Abbiamo bisogno di attivare attraverso il Fondo di solidarietà nazionale - è stato fatto per la Regione Sicilia

È un dramma che va superato e questo sforzo è stato fatto attraverso questo provvedimento. Qui voglio ringraziare il ministro Lollobrigida e tutta la sua struttura per l'impegno, il sottosegretario La Pietra, che ringrazio per la sua disponibilità,

sono stati presentati 863 emendamenti, li abbiamo analizzati tutti per arrivare ad approvare 77 emendamenti e 14 ordini del giorno. Questo contributo del Parlamento, dei senatori e delle senatrici è fondamentale, che sollevavano temi che non è stato possibile inserire, sicuramente faranno da *database* per la Commissione per sviluppare altri provvedimenti importanti. Oggi esprimiamo quindi, come Gruppo Lega-Salvini Premier,

leggere la nota dei nostri uffici legislativi per vedere che in questo provvedimento ci sono decine di misure a favore dell'agricoltura e dei nostri agricoltori. *(Applausi)*. Continuiamo a difendere gli agricoltori, presidio del territorio

atmosferici che hanno colpito il nostro Paese, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. In Val d'Aosta abbiamo visto i disastri di questi ultimi giorni, che fanno il paio con la siccità della Sicilia, che vengono dopo gli eventi alluvionali della Toscana,

che i cambiamenti climatici esistono, perché in quest'Aula non sempre da parte di chi governa c'è stato un riconoscimento del fatto che c'è un cambiamento climatico in atto e che di pari passo è necessario che siano fatte anche politiche volte a prevenire questi fenomeni. È chiaro che sono fenomeni rispetto ai quali non possiamo decidere singolarmente, ma non possiamo nemmeno pensare che o si fa tutti insieme o non si fa nulla. Bisogna cioè intervenire sulle infrastrutture, bisogna essere preparati

che sono necessari (si è parlato dei ristori in vari settori), ma è anche chiaro che una serie di ristori deriva da una mancata gestione di problematiche che sono presenti, sono a carico dei nostri agricoltori, ma non sono state né contenute né risolte anche in questi ultimi due anni. Lo abbiamo detto ieri sul tema del granchio blu, rispetto al quale la situazione in questi ultimi due anni è gravemente peggiorata, o sul tema della

ex ministri Centinaio, Patuanelli e gli altri che si sono susseguiti. E sentir dire sempre in quest'Aula che quelli che c'erano prima non hanno fatto niente e che sono bravi solo quelli che gestiscono ora mi sembra mortificante per tutti quelli che hanno lavorato al servizio del Paese. Mi sembra poi altrettanto mortificante per tutti quegli agricoltori che nel Dopoguerra avevano un Paese e dei poderi in rovina e che si sono fatti i calli alle mani ristrutturando i poderi, impiantando i vigneti, portandoli in giro per il mondo ed inventando il *made in Italy,* che non è stato creato in questi due Oggi parliamo di *made in Italy* perché dal dopoguerra (e anche da prima) ad oggi sono state fatte politiche di un certo tipo, che non sono state inventate in questi due anni. Oggi si parla di mancata redditività delle aziende, di crisi del mercato, di epidemie, si parla di problemi, forse anche perché in questi ultimi due anni non si è fatto a sufficienza per lenirli e forse perché quella redditività che le aziende hanno avuto per tanti anni con tante difficoltà oggi è venuta meno. Allora poniamoci un problema: forse sarebbe meglio

Anche in questo decreto-legge il confronto è stato pari a zero. Questo non perché la Commissione ha voluto che non ci fosse (devo infatti ringraziare il Presidente, i commissari, i relatori e il Sottosegretario), ma perché i decreti-legge strozzano la democrazia parlamentare, non consentono di affrontare i problemi in profondità, non consentono di intervenire in quei punti normativi che avrebbero bisogno di piccoli o grandi interventi per migliorarli, non nell'interesse della parte politica che governa, ma nell'interesse del Paese. Questo è uno dei temi. collega con esperienza parlamentare era che quando si parla spesso non si viene ascoltati. Questo sta avvenendo anche ora e mi dispiace anche che non mi ascolti nemmeno il Presidente della 9a Commissione,

cioè che non sarà consumato un metro quadrato di suolo. Egli ci ha dato tutta un'illustrazione; ebbene, fra qualche mese, fra qualche anno andremo a prendere quello che si è dichiarato e lo constateremo con i fatti, sperando di essere smentiti, perché se l'agricoltura cresce, progredisce, prosegue nel suo percorso di questi anni, noi siamo contenti, perché il settore primario ha avuto le sue giuste soddisfazioni ed un bene nell'interesse del Paese. Come ho detto ieri,

dobbiamo dire che il direttore di Agea, venuto in audizione il 3 aprile scorso, non ci ha detto niente di quello che avveniva e ci siamo trovati sul tavolo la riorganizzazione di un'agenzia che eroga quattro miliardi di contributi alle aziende agricole che sono vitali per pagare anche i mutui. Infatti, è inutile fare

le aziende piccole che presidiano il territorio e che sono essenziali e le grandi aziende. Esse sono funzionali le une alle altre. Il sistema funziona se la produzione dialoga con la trasformazione, se le piccole aziende dialogano con le grandi, se il sistema di gestione faunistico-venatorio (cioè il mondo dei cacciatori) dialoga con l'agricoltura e l'agricoltura dialoga con l'ambiente e viceversa. Diversamente, il sistema va in crisi. E se si pensa che un settore possa agire autonomamente, commettiamo un grande errore perché l'agricoltura è un sistema produttivo che ha molti più aspetti di tanti altri settori. Tra questi, ci sono la gestione faunistico-venatoria, l'ambiente e il mercato.

Il provvedimento tocca punti fondamentali per sostenere le nostre imprese impegnate in un settore particolarmente provato da fattori climatici avversi e dalla situazione internazionale che, per esempio, nel caso dei produttori di grano duro, alla luce delle recenti crisi sanitarie, nonché della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, hanno comportato e stanno comportando ancora una forte sofferenza della filiera. Non mancano misure per il contrasto della peste suina che mette a dura prova un settore di eccellenza apprezzato in tutto il mondo per la qualità e la bontà dei nostri prodotti. Per affrontare con più incisività la questione abbiamo previsto l'aumento dei poteri del Commissario. poi misure tese a evitare il consumo di suolo coltivabile a vantaggio dell'agrivoltaico (e lo facciamo senza andare a toccare i progetti già avviati o quelli di diretta derivazione del PNRR). Abbiamo stanziato ingenti risorse per il contrasto alla peronospora e alla xylella, prevedendo anche la nomina di un commissario, e per il contrasto al granchio blu. Prevediamo misure di contrasto alle pratiche sleali, con l'introduzione della nozione di costo medio di produzione. La pratica sleale falsa il mercato a discapito della sicurezza dei lavoratori e della qualità del prodotto. Non da ultimo, cosa di cui sono orgoglioso, visti anche gli ultimi episodi di cronaca, è stata introdotta la misura tesa a combattere quell'infame pratica, troppo spesso presente in alcune realtà, che è il caporalato *(Applausi)*, grazie agli emendamenti del relatore, presidente De Carlo, all'articolo 2. Era giusto che ci occupassimo anche della grave situazione connessa alla scarsità idrica, di assicurare continuità operativa all'ex Ilva e di supportare le imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale. Per deformazione professionale sono portato come sempre a guardare i numeri per capire quanto importante ed incisivo sia il settore nell'ambito economico nazionale. Ebbene, il valore del sistema agroalimentare italiano complessivamente si aggira ai 621 miliardi di euro di fatturato, il 15 per cento del PIL nazionale, confermandosi un pilastro economico del nostro Paese. Per quanto riguarda l'*export*, nel 2023 il settore agroalimentare italiano ha raggiunto la quota di 64 miliardi di euro: risultato storico mai raggiunto prima, in aumento di circa il 6 per cento rispetto all'analogo dato del 2022. Il dato è destinato ad aumentare se, come già da tempo sta facendo questo Governo, si contrasta il fenomeno dell'*italian sounding*, che oggi è stimato in un valore di oltre 100 miliardi di euro, e promuovendo sempre con forza il nostro *made in Italy*. Sono 100 miliardi di euro quelli spesi sul mercato estero da consumatori che pensano di comprare prodotti italiani, ma che invece di italiano hanno solo un'assonanza, cioè il *sounding*, che richiama il nome italiano, senza la qualità e la sicurezza che contraddistinguono i nostri prodotti. Ricordo solo il vitivinicolo, come esempio del *made in Italy*, che vale 45 miliardi ed è un'eccellenza riconosciuta a livello mondiale. Dal punto di vista occupazionale, con oltre 1,5 milioni di lavoratori impiegati nel 2022, il settore si colloca al 7 per cento del totale di tutto il mondo lavorativo nazionale, in controtendenza rispetto ad altri settori. L'Italia si conferma al primo posto per numero di riconoscimenti conferiti dall'Unione europea: tra il 2020 e il 2021 questi passano da 312 a 315, inclusi DOP, IGP e STG. Vorrei anche ricordare che proprio lo scorso maggio è stato sottoscritto un accordo tra il Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e forestale e Cassa depositi e prestiti, con la collaborazione di un'importante banca italiana, per rendere nuovamente competitivo uno dei comparti che nobilita maggiormente l'industria italiana, incidendo in maniera importante sul PIL nazionale. Alla base dell'accordo c'è la volontà di promuovere politiche creditizie e sinergie destinate allo sviluppo del sistema agricolo rurale e agroalimentare, potendo anche attingere a risorse del PNRR. Il programma prevede un'azione congiunta per investimenti destinati a filiere agroalimentari, ricerca, innovazione, accesso ai mercati esteri, maggiore efficienza per il risparmio energetico, più attenzione all'economia circolare e al passaggio generazionale, che ha da sempre rappresentato una delle maggiori sfide per l'agricoltura europea, in particolare per quella italiana. In particolare, la strategia per i giovani e il ricambio generazionale saranno realizzati in maniera diretta attraverso il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e l'intervento di sviluppo rurale per l'insediamento dei giovani nelle nostre imprese agricole. Il fine è quello di offrire uno strumento per attrarre i giovani nel settore agricolo e per consentire di attuare le loro idee imprenditoriali, il tutto da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2027. Questo a testimoniare, ove ve ne fosse ulteriore bisogno, l'attenzione che il Governo sta dando all'intero comparto, puntando fortemente sul rilancio e sullo sviluppo. Tornando al decreto, è evidente che sono tanti i temi del settore toccati dal provvedimento, che è stato lungamente oggetto di discussione in Commissione. A tal proposito, consentitemi di ringraziare i relatori, il presidente De Carlo e il senatore Bergesio. I temi sono tanti, perché ancora una volta il Governo Meloni deve affrontare e risolvere problemi che erano giacenti a causa del poco dinamismo dei Governi precedenti. Non per aprire polemiche, ma da due anni a questa parte è invalsa in quest'Aula la deprimente pratica di criticare a prescindere l'operato del Governo, senza fornire nessuna valida alternativa se non demagogiche quanto inapplicabili proposte che ci portano a fare una sola domanda: dove eravate fino a due anni fa? Allora, Presidente, è fisiologico che la gente lì fuori, con la quale non abbiamo mai perso il contatto, a differenza di altri, perché rivendichiamo con forza la nostra appartenenza al popolo, ci premi quando si tratta di andare alle urne e di esprimere una preferenza. Il popolo ci premia perché abbiamo presentato un programma e lo stiamo portando avanti con coerenza. La coerenza è il tratto distintivo di questo Governo. Quello che abbiamo detto che avremmo fatto lo stiamo in effetti facendo, con buona pace di chi, uscito precedentemente precedentemente perdente dalle urne, oggi rivendica soluzioni miracolose che, non si sa perché, non ha attuato quando aveva la forza e i numeri per farlo. Scusi lo sfogo, Presidente, ma sono anche stanco di essere additato come sostenitore di un Governo antidemocratico, quando è stata proprio la democrazia, con i suoi meccanismi condivisi e accettati, che ci ha dato la possibilità di portare avanti un programma annunciato agli elettori prima delle elezioni, premiato dagli stessi come valido e che oggi abbiamo la sola colpa di attuare come promesso in campagna elettorale. Pertanto, signor Presidente, ringraziando anche il ministro Lollobrigida e il sottosegretario La Pietra per l'impegno profuso, con l'orgoglio per l'appartenenza a questo Gruppo parlamentare, annuncio il voto favorevole di Fratelli d'Italia al provvedimento in esame.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

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per le disabilità. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, considerata la diretta televisiva in corso.

Nessy Guerra, cittadina italiana di 25 anni, è stata arrestata in Egitto e posta sotto processo dopo le accuse di adulterio avanzate dal marito italo-egiziano, dal quale si sta separando, rischiando così due anni di carcere e di perdere la custodia della figlia: in Italia, l'uomo è stato condannato in via definitiva per violenza sessuale, stalking e lesioni verso la precedente compagna, ma il consolato egiziano di Milano non ha trasmesso al tribunale il certificato di condanna, pur essendo stato questo tradotto; gli avvocati egiziani che assistono Nessy Guerra hanno nel frattempo presentato appello e convinto sua madre a convertirsi all'Islam, con la speranza che, concluso il processo per adulterio, la figlia possa essere almeno affidata alla nonna materna, la quale si trova attualmente con la figlia e la nipote in una località segreta dopo le costanti e violenti minacce ricevute dal marito; gli avvocati difensori hanno ribadito più volte la fondamentale importanza, per le sorti del processo, del certificato di condanna del marito di Nessy Guerra, attualmente fermo nel consolato egiziano di Milano, il quale consentirebbe una svolta nel processo e aumenterebbe la possibilità che la figlia venga affidata alla donna italiana o in alternativa alla nonna materna, gettando luce sulla capacità vessatoria e la natura violenta del marito; organi di stampa riferiscono di uno sconcertante e assoluto disinteresse del consolato italiano in Egitto e del Ministro in indirizzo, nonostante i numerosi solleciti della famiglia e dei difensori di Nessy Guerra, di assoluta urgenza che le autorità diplomatiche italiane si attivino rapidamente instaurando appositi canali con le autorità egiziane per sbloccare al più presto l'invio del casellario penale del marito di Nessy Guerra verso il tribunale di Hurghada, al fine di fornire una essenziale prova nel processo. Signor Ministro, io ho riferito notizie degli organi di stampa, mi auguro però e spero moltissimo di essere smentita. pertanto di sapere quali siano le condizioni di Nessy Guerra e di capire quali sono le azioni che intende adottare per sollecitare la trasmissione di questo certificato e scongiurare l'ipotesi che la figlia

È necessario quindi che il Governo faccia la propria parte e si attivi in modo tempestivo. Le chiediamo, quindi, di sapere che cosa state facendo, con quali iniziative e con quali tempistiche.

abbiamo seguito fin dall'inizio il caso della signora Nessy Guerra e della piccola Aisha. È una vicenda che ci sta molto a cuore, come ho ribadito molto chiaramente anche al nuovo ministro degli esteri egiziano Abdelatty, nominato ieri sera, in una lettera che gli ho appena inviato. La nostra ambasciata mantiene costanti contatti con la connazionale, con i familiari e i suoi legali. Al momento la signora Guerra si trova in Egitto con la bambina ed entrambe sono in buone condizioni di salute. La signora Guerra infatti non è più in stato di detenzione: era stata arrestata il 12 aprile a seguito della denuncia di adulterio presentata dal marito, ma è stata rilasciata due giorni dopo anche grazie all'immediato intervento della nostra ambasciata. La bambina, essendo anche cittadina egiziana, non può lasciare il Paese senza il consenso di entrambi i genitori. Sul punto l'ambasciata sta intraprendendo ogni possibile iniziativa anche in qualità di giudice tutelare per giungere a una soluzione condivisa. Sul piano legale la connazionale ha nominato un avvocato e promosso un giudizio *in loco* per ottenere l'affido della bambina. Lo scorso 26 giugno il tribunale della famiglia egiziana ha emesso la sentenza di primo grado e ha deciso di non concedere l'affidamento alla madre. In vista del giudizio d'appello, l'avvocato ha chiesto di acquisire e legalizzare il casellario giudiziale del marito della signora Guerra. Abbiamo prontamente sensibilizzato il consolato generale egiziano a Milano e la documentazione legalizzata è ora disponibile. L'ambasciata ne ha dato pronta comunicazione al legale italiano della signora Guerra ai fini della trasmissione alle competenti autorità egiziane. Come facciamo su ogni caso che riguardi i minori, abbiamo dato massima priorità alla questione, assicurando ogni possibile assistenza alla signora Guerra e alla piccola Aisha. Continueremo a lavorare per difendere la dignità e i diritti delle nostre nostre due concittadine. Lo faremo con le strutture del nostro Ministero, con serietà e riservatezza. Il nostro obiettivo è giungere a una soluzione positiva e rapida della vicenda nel superiore interesse della minore. Continueremo al contempo a tenere alta l'attenzione politica su questo caso nei nostri contatti con le autorità governative egiziane. la ringrazio. È diventata purtroppo ormai una abitudine per noi vederci in questa situazione per parlare di italiani all'estero. Abbiamo avuto il caso Salis, quelli di Filippo Mosca in Romania e Matteo Falcinelli in Florida e adesso il caso di Nessy Guerra. Ho ascoltato volentieri la sua risposta, conosco la professionalità e l'operosità dei nostri diplomatici e so che sia quelli a Roma che quelli nella rete diplomatica e consolare si danno da fare al massimo delle loro possibilità. Chiederei però a lei di avere un atteggiamento anche in questo caso un po' meno felpato di quello che ci ha illustrato nei casi precedenti. Sono infatti un po' preoccupato del fatto che i nostri connazionali riescano ad avere l'attenzione del Ministero soltanto quando il loro caso finisce sui giornali. Sempre più spesso accade e, se accade, è perché c'è evidentemente una percezione del fatto

alla fine hanno anche ragione. Lei diceva che Salis farebbe meglio a star zitto. Ma, dal punto di vista di Roberto Salis, sua figlia è uscita di prigione proprio proprio grazie al rumore che ha fatto, al contrario dei consigli che ha ricevuto. È chiaro che normalmente se si lascia lavorare il Governo nel silenzio, questo può agevolare i contatti diplomatici. Se però poi i risultati non arrivano, capisco che i nostri concittadini ricorrano alla stampa. Anche nel caso di Nessy Guerra, quindi, continueremo a seguire la vicenda. La preghiamo di farsi sentire e di alzare anche un po' la voce, perché il tono felpato va bene, ma, se poi diventa un sopire, troncare di manzoniana memoria, è evidente che non portiamo i risultati a casa.

Gentile Ministro - come già si è detto - so che lei ha presenziato lunedì alla importante inaugurazione della divisione centrale del tribunale unificato dei brevetti di Milano, che affiancherà le divisioni di Parigi e Monaco di Baviera e avrà competenza sui contenziosi relativi ai settori medicale-farmaceutico, agroalimentare, fitosanitario e moda, settori davvero importanti per il nostro Paese. L'assegnazione di una delle divisioni centrali del TUB è un riconoscimento all'Italia quale seconda economia manifatturiera d'Europa e mette Milano, la città che lo ospita, sempre più al centro del nuovo sistema europeo di protezione della proprietà intellettuale, strumento essenziale per tutelare la competitività delle imprese italiane sui mercati esteri. Il risultato è stato ottenuto al termine di un complesso negoziato a livello europeo, in cui il nostro Paese è stato in grado di ottenere questo importante risultato. E non va dimenticato che l'avvio a pieno regime del nuovo sistema brevettuale unificato coincide con l'inizio di una nuova legislatura europea. Anche questo contesto ci deve far riflettere. Ora l'Unione è chiamata a dotarsi di una politica industriale ambiziosa e pragmatica, in grado di rilanciare la competitività e far fronte alle nuove sfide per i settori produttivi. Pensiamo ai rischi geopolitici, alla diversificazione dei mercati di approvvigionamento e di sblocco, all'innovazione tecnologica e ai cambiamenti climatici. Le chiediamo, signor Ministro, quali ricadute potrà generare effettivamente il nuovo polo giurisdizionale di Milano sulle imprese, sugli operatori del diritto nel settore della proprietà industriale,

Signora Presidente, la nuova sede del tribunale unificato dei brevetti è un risultato dal grande significato politico per l'Italia in ambito europeo: un successo importante anche perché ottenuto al termine di quello che considero un esempio di negoziato europeo virtuoso; un negoziato che il Governo ha condotto con pazienza e pragmatismo. Abbiamo lavorato tutti insieme, a differenza di altre iniziative in passato - Governo, Regione, Comune, magistratura ed esperti - e abbiamo avuto come unica stella polare l'interesse nazionale. Il risultato ottenuto è tangibile e non era affatto scontato, e per questo voglio anche ringraziare i diplomatici e i funzionari della nostra rappresentanza diplomatica presso l'Unione europea. È con il gioco di squadra e con un approccio concreto e non ideologico che si ottengono i risultati in Europa. Avere in Italia la sede del tribunale unificato dei brevetti è una scelta europeista che fa sempre più di Milano una delle capitali europee dell'innovazione. Le competenze della divisione centrale di Milano riguardano settori chiave del sistema industriale italiano. Penso al settore farmaceutico, alla moda, al *design*, al fitosanitario e all'agroalimentare: tutti ambiti in cui il saper fare italiano è motore di innovazione, e lo dimostrano i numeri in evidente crescita. L'Italia è al terzo posto per domande di brevetto europeo. Nel 2023 le richieste italiane di brevetti, anche nei settori tecnologici di punta, sono state superiori alla media europea. Grazie alla giurisdizione unificata, le nostre imprese potranno ora tutelare i propri investimenti e brevetti senza dover affrontare procedimenti paralleli in diversi Paesi. La certezza delle regole è d'altronde il migliore strumento per attirare investimenti stranieri in Italia e sostenere le nostre esportazioni, che sono in costante aumento; merito del dinamismo delle nostre aziende, il cui *export* il cui *export* vogliamo rafforzare anche con la diplomazia della crescita che ho messo in atto fin dall'inizio del mio mandato. A dicembre organizzeremo a Milano gli stati generali dell'*export* e li faremo coincidere con la conferenza degli ambasciatori italiani nel mondo. Anche a livello europeo la competitività deve essere una priorità assoluta, insieme a una politica industriale che metta al centro le imprese e le metta nella condizione di investire e innovare. Nella nuova legislatura europea vogliamo creare un ambiente sempre più favorevole agli investimenti e per questo serve un quadro normativo chiaro e semplificato, che non gravi sulle imprese e tuteli i lavoratori. Il nostro approccio è sempre stato chiaro: portare l'Unione europea su posizioni pragmatiche e non ideologiche, lontane dagli estremismi e più vicine ai bisogni dell'economia reale e dei cittadini. L'Italia in Europa ha molte cose da dire e da dare. Andiamo avanti sulla scia di un successo come quello del tribunale dei brevetti.

per favorire la competitività delle nostre imprese. E questo tanto più alla luce del *boom* che c'è stato nel 2023: si registrano, infatti, 5.053 nuove domande di brevetti ed è un nuovo *record* per l'Italia. È quindi un bene che si guardi all'internazionalizzazione delle nostre imprese

di cui molti sono giovani. È un'emigrazione atomizzata, non come quella di un tempo quando si muovevano intere comunità, magari alla ricerca di un nuovo destino nel nuovo mondo; in questo caso, spesso, si tratta invece di gente formata, di cervelli, di risorse reali che perdiamo.

ci sono Paesi sui quali in sede bilaterale (per esempio Spagna e Francia) è stata ammessa la doppia cittadinanza. abbia *in itinere* un accordo da concludere con la Spagna - mi auguro presto, e sono queste le notizie che chiedo di fornirci al signor Ministro - per consentire la doppia cittadinanza e, quindi, il mantenimento per i cittadini italiani della loro cittadinanza. È un fatto che ritengo interessi tutti noi e il sistema Italia.

Signora Presidente, Italia e Spagna sono legate da relazioni particolarmente strette, relazioni tra popoli prima ancora che fra Stati e Governi. La comunità italiana residente in Spagna e quella spagnola in Italia contribuiscono significativamente alla vita economica, sociale e culturale dei due Paesi. La nostra presenza in Spagna è particolarmente significativa, avendo ormai superato le 300.000 unità: è praticamente triplicata nell'ultimo quindicennio. Parliamo - come diceva lei - di un'immigrazione nuova, giovane, qualificata, che si sente europea. Sin dall'inizio del mio mandato mi sono concentrato sull'efficienza della nostra rete consolare, sulla quantità e qualità dei servizi ai nostri connazionali, in particolare nei Paesi con importanti e crescenti comunità italiane, come appunto la Spagna. Anche per questo ho deciso di riaprire il consolato generale d'Italia a Madrid, che è operativo dallo scorso lunedì. Sappiamo che molti italiani residenti in Spagna vorrebbero poter acquisire la cittadinanza spagnola, senza però dover rinunciare a quella italiana. Diversamente dalla legge italiana - come lei ricordava - quella spagnola impedisce la doppia cittadinanza. Le uniche eccezioni alla regola in ambito europeo valgono per i tre Paesi confinanti, Francia e Portogallo ed Andorra. Per venire incontro alle aspettative della nostra collettività, abbiamo proposto al Governo spagnolo di siglare un accordo bilaterale in materia. Le autorità di Madrid hanno avviato le procedure interne per la revisione del testo, in un periodo che è però coinciso con le elezioni parlamentari anticipate e la successiva articolata formazione del nuovo Governo Governo a Madrid. Abbiamo letto con favore le parole del ministro degli esteri Albares sull'accordo. Confidiamo ora che il Governo spagnolo passi dalle parole ai fatti. Contiamo quindi sull'impegno fattivo del Governo di Madrid per finalizzare l'intesa quanto prima, nell'interesse dei nostri connazionali che sono ormai pienamente integrati in Spagna.

Governo spagnolo, ma era giusto che arrivassero rassicurazioni e, se me lo permette, le chiederò qualcosa in più. Il tema che ho citato è più vasto - è una

per poter lavorare laddove erano andati. Pur avendo acquisito un'altra cittadinanza, si sentono legati al nostro Paese, sono italiani come noi, hanno la nostra formazione, i nostri valori spirituali, culturali, parlano la nostra lingua.

*(M5S)*. Signor Ministro, nel 2019 il Comitato olimpico internazionale ha assegnato alle città di Milano e di Cortina l'organizzazione dei Giochi olimpici invernali del 2026. Nel *dossier* di candidatura si legge che il piano complessivo di realizzazione dei giochi prevedrà una valutazione ambientale strategica complessiva (VAS), che sarà condotta da una commissione *ad hoc*, e sarà inoltre sottoposto ad una specifica valutazione per evitare ogni possibile impatto sulla conservazione della biodiversità e e del patrimonio culturale, al fine di garantire che si tengano in conto dei fattori ambientali in sede di sviluppo delle azioni strategiche. Le autorità coinvolte dovranno stabilire se i progetti dovranno essere preliminarmente sottoposti a una valutazione di impatto ambientale (VIA) specifica, sotto la responsabilità delle Regioni. Già l'allora Ministro della transizione ecologica aveva informato che, tra i diversi interventi previsti all'interno di siti della rete Natura 2000, alcuni hanno comportato o comporteranno la necessità di attuare la procedura di deroga prevista dalla direttiva *habitat*, a seguito di valutazione di incidenza conclusa con esito negativo, e che il Ministro stava curando la trasmissione alla Commissione europea delle misure di compensazione. Va considerato che il piano degli interventi interessa l'intera regione alpina; che le Dolomiti dal 2009 sono patrimonio Unesco; che la nuova pista da bob, che si è deciso di iniziare a costruire a Cortina nonostante il parere contrario dello stesso CIO, occupa un intero crinale della conca d'Ampezzo, che è uno dei più importanti contesti montani al mondo, interamente sottoposto a vincolo paesaggistico; che il progetto non è stato sottoposto alla valutazione di impatto ambientale prevista dalla direttiva del 2011, nonostante l'infrastruttura abbia un impatto ambientale, idrogeologico, forestale, paesaggistico ed ecosistemico significativo; che per la realizzazione della pista è stata tagliata una foresta di larici secolari di 20.000 metri quadrati, senza alcuna valutazione ambientale, nonostante il taglio degli alberi sia una delle attività elencate nell'allegato 2 della direttiva. Nelle Regioni coinvolte sono diverse le opere da realizzare o su cui insistono i progetti di ristrutturazione. In Lombardia, per esempio, si pensi ai villaggi olimpici: quello di Milano impermeabilizza il 90 per cento dei 250.000 metri quadri dell'intera superficie; o, sempre a Milano, il PalaItalia Santa Giulia, il palazzetto destinato ad ospitare le gare di hockey maschile, per il quale nel gennaio del 2019 il *dossier* dava atto della necessità della preliminare pubblicazione della valutazione ambientale strategica. Tuttavia, nel decreto del Presidente del Consiglio del 2022 si afferma che il piano degli interventi rileva quale programma finanziario non assoggettato alla procedura di valutazione ambientale strategica e quindi approva il piano predisposto dalla Simico senza alcuna indicazione Anche il piano complessivo delle opere olimpiche, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio nel settembre del 2023, non è stato sottoposto alla valutazione ambientale prevista dalla direttiva, che viceversa la procedura di VAS deve essere effettuata su piani e programmi che possano avere significativi impatti sull'ambiente. Si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda procedere alle valutazioni ambientali omesse, prima della completa realizzazione delle opere olimpiche, in ossequio alle direttive europee e alla legislazione nazionale di settore;

e la Fondazione Milano-Cortina 2026, tutti gli aspetti relativi alle valutazioni ambientali connesse alle opere relative ai Giochi olimpici. Dall'esame della documentazione fornita dalla predetta società, si è rilevato che alcune opere rientravano nell'ambito della pianificazione di settore e degli strumenti urbanistici già vigenti. Pertanto non era necessario lo svolgimento di un'ulteriore e autonoma valutazione ambientale strategica Resta fermo che, qualora le opere costituiscano variante, i relativi piani di riferimento debbano essere sottoposti a VAS. Invece, alcuni degli interventi sono sottoposti a VIA o a verifiche di assoggettabilità, nonché a valutazione di incidenza ambientale in presenza di interferenze con i siti della rete Natura 2000, che lei ha citato. In ogni caso, nell'espletamento delle varie procedure di valutazione è stata evidenziata la necessità di garantire per tutti gli interventi la valutazione degli effetti cumulativi derivanti dall'insieme delle progettualità che insistono sullo specifico territorio. in relazione al programma di realizzazione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, è prevista una procedura di VAS complessiva per l'intero territorio interessato dai giochi, sulla base di un protocollo d'intesa tra le Regioni e le Province autonome interessate. Le valutazioni ambientali dovranno svolgersi nel rispetto della normativa nazionale ed euro-unitaria. Per quanto concerne la nomina dei membri della nuova commissione VIA-VAS, ad oggi sono stati nominati 41 componenti sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute; le restanti nomine sono in corso di perfezionamento e garantiranno il giusto equilibrio tra le diverse professionalità richieste per la commissione, oltre che quelle di genere. È mia intenzione procedere rapidamente alla nomina degli ulteriori componenti per garantire il *plenum* della commissione, la cui operatività è sempre stata garantita anche in questa breve fase di transizione, perché comunque era in *prorogatio* e continuava ad operare.

nel senso che non esiste un elenco esaustivo delle opere, sia stabili, sia temporanee, legate all'iniziativa, registrando di fatto mancanza di comunicazione, pubblicità e trasparenza. Apparirebbe opportuno, a questo punto, quantomeno la realizzazione di un portale unico della trasparenza dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, che dia la possibilità di individuare tutte le opere sia di competenza della Fondazione sia della Simico sia di Anas, di monitorare passaggi e l'*iter* delle opere, sia stabili che temporanee, le spese relative all'organizzazione, alla promozione dei giochi, oltre alle valutazioni di impatto ambientali con dati disaggregati in formato aperto. Di fatto, si sta intervenendo su un territorio già molto fragile e si sta intervenendo senza una valutazione preventiva dell'effetto cumulativo degli interventi che vengono posti in essere. Penso semplicemente al fatto di aver privilegiato i collegamenti via strada invece di quelli via ferro. Non si è fatto il collegamento dall'aeroporto Orio al Serio, non si sono collegate le città di Cortina e di Bormio con un trenino, magari anche carino dal punto di vista turistico. Si sono costruite strade, si è consumato suolo. L'impatto ambientale è altissimo, ma ciò non risulta da nessuna parte, come non risultano le misure di compensazione dovute.

Signor Presidente, il Gruppo del Partito Democratico interroga il Ministro e, per suo tramite, il Governo, su quella che chiamare emergenza diventa ormai un termine desueto, perché è una urgenza che è emersa. Ieri «Il Sole 24 ore» Sole 24 ore» in prima pagina evidenziava questo disastro ambientale in corso. Noi non abbiamo soltanto una Italia spaccata dalle iniziative legislative di questo Governo, ma ormai spaccata anche dal punto di vista dell'urgenza climatica.

insostenibile. In questo momento, in Sicilia, più di cento Comuni hanno l'interruzione della fornitura di acqua potabile. potabile. Il lago di Pergusa, un luogo storico raccontato anche dalla nostra letteratura antica, si è prosciugato: un ecosistema distrutto e urgenza dal punto di vista del turismo. Nella Sicilia orientale, abbiamo raggiunto un livello di precipitazioni, negli ultimi sei mesi, inferiore a quello che già vi era stato, più di dieci anni fa, con la crisi climatica e idrica della Sicilia. Sono state fatte diverse iniziative, anche dai Governi precedenti, che hanno impostato il tema della siccità sul piano nazionale, in alcuni casi con un piano, Italia Sicura. Niente è stato fatto in particolare nella Sicilia. negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, persino l'associazione che raggruppa diversi centri di dialisi ha lanciato l'allarme per la carenza dell'acqua. È un tema che riguarda tutto il Mezzogiorno, ma il punto fondamentale è che i dati pubblicati sembrano non interessare il Governo. Quindi, la prima cosa che noi chiediamo a lei, signor Ministro, e al Governo, è se siete a conoscenza di questi dati, se siete a conoscenza del fatto che non si parla ormai soltanto di emergenza, ma di vera e propria desertificazione. I danni che sono stati calcolati, per esempio in Sicilia, raggiungono ormai i due miliardi. Abbiamo intere parti del territorio agricolo desertificate, con una crisi irreversibile anche nel settore della zootecnia. A fronte di questo, tutta una serie di attività, che pure erano state promesse dal Commissario che voi avete nominato, non sono state realizzate. Da questo punto di vista, la nostra richiesta è, innanzitutto, se siete a conoscenza di questi dati. Poi, di sapere che cosa avete fatto fino a questo momento, ma soprattutto se non ritenete che sia necessaria, per quanto ormai tardiva, una cabina di regia di tutto il Governo con il Commissario per cercare di capire come fare, a partire da quei fondi PNRR che avete spostato, soprattutto per il Sud, sul Fondo di sviluppo e coesione. Stiamo parlando di diversi miliardi che non hanno trovato applicazione, così come su tutta la parte che riguarda il dissesto idrogeologico. Noi possiamo semplicemente dare voce alle tante persone che in questo momento vivono una disperazione, non soltanto per le proprie attività agricole del momento e i danni che subiscono, ma perché vedono e sono consapevoli del fatto che c'è una irreversibilità che si è mantenuta. Quindi, da questo punto di vista siamo già in una zona di danno, non di ricostituzione di ciò che c'era prima. Ci chiediamo a questo punto perché questo Governo, che pure ha nominato un ministro della siccità che per ironia della sorte si chiama Dell'Acqua, ritenga che noi si debba avere non soltanto un'autonomia differenziata, ma anche un'autonomia

Grazie, Presidente, e grazie agli interroganti. In merito ai quesiti posti, lo scorso 6 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, per la durata di dodici in relazione alla situazione di grave *deficit* idrico in atto nel territorio siciliano. Per l'attuazione dei primi interventi sono stati stanziati 20 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali. Il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato, con successiva ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, commissario delegato per la realizzazione degli interventi urgenti, attraverso la predisposizione di un piano che deve garantire *in primis* *in primis* l'approvvigionamento idropotabile della popolazione. Il piano può essere chiaramente rimodulato ed integrato, anche con ulteriori risorse finanziarie, sulla base della necessità di finalizzare o ampliare le misure previste. Lo scorso 7 giugno è stato approvato il piano degli interventi, comprensivo di 138 attività, per un importo complessivo pari ai 20 milioni di euro già stanziati, più 1 milione e 200.000 euro a valere sulle risorse regionali. Il Dipartimento della protezione civile segnala che, a seguito di interlocuzione con il commissario delegato, sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare la necessità di azioni aggiuntive per fronteggiare l'emergenza in atto. Per quanto attiene alle altre Regioni meridionali, si segnala che attualmente nelle Regioni Basilicata e Calabria vi sono alcune zone classificate in criticità con grado di severità media, connessa al mancato soddisfacimento dei fabbisogni idrici. Siamo in fase di valutazione degli effetti di "medicazione" delle azioni poste in essere. In ogni caso, allo stato attuale non sono comunque pervenute richieste di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale. Accanto alle ordinarie competenze attribuite al MASE in materia di prevenzione dei fenomeni siccitosi, si ricordano le azioni messe in atto sin dallo scorso anno con il decreto-legge siccità, contenente una serie di misure utili ad incrementare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e la riduzione della dispersione di risorse idriche, anche attraverso la nomina del Commissario straordinario nazionale, che si avvale, nella propria azione, dei dati forniti dagli osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici istituiti presso ciascuna Autorità di bacino. Lei ha detto che l'Italia è spaccata dalle iniziative del Governo. La realtà è antica, mi permetta. Ahimè, abbiamo 2.391 gestori del servizio idrico. Proprio in Sicilia c'è ancora la situazione di maggiore difficoltà nel creare l'accorpamento, per ragioni locali. L'ultima rimasta è la Provincia di Trapani, in questo caso. Stiamo andando avanti spingendo le realtà, proprio per arrivare a ridurre quei 2.391 gestori, che è il disegno nazionale che ha passato tre Governi (quindi non è da accreditare a questo Governo), a una

di perdite sul sistema idrico e ci crea difficoltà su questo sistema. Naturalmente queste sono poi le conseguenze di interventi che sono sempre di emergenza e invece non dovrebbero essere di emergenza. Al di là del cambiamento climatico, che non è imputabile al Governo, in questo caso rispetto alla siccità.

per 140 interventi, significa assicurare poche decine di migliaia di euro per ogni intervento. D'altra parte lei, per la posizione che riveste, cioè quella di Ministro dell'ambiente, si rende conto che qui non siamo di fronte ad un evento, ma ad un fenomeno, che viene annunciato da tendenze che sono misurate ormai da anni. Quindi non si può pensare che si scopre l'emergenza il 6 maggio, e il 7 giugno si fa qualcosa tra cui, tra l'altro, dare soltanto 20 milioni rispetto ad una questione che ha già superato i 2 miliardi di danni solo in Sicilia, per non parlare delle altre Regioni d'Italia. In realtà questo ritardo è dovuto sia all'inerzia del Governo sia, in fondo, all'eco di un forte negazionismo climatico che solo questo Governo ha, che si misura adesso con la consapevolezza dei danni e che produce questo effetto. Non credere al fatto che non piove significa semplicemente non rendersi conto non soltanto delle esigenze che ci sono oggi, ma soprattutto di quelle che riguardano le generazioni future. La Sicilia in questo momento è assetata, come la Sardegna, la Calabria, la Campania, la Basilicata. C'è un Sud che non ha ricevuto attenzione e che nei prossimi mesi vivrà situazioni ancora più drammatiche. Non è possibile avere avere questo tipo di risposte né tantomeno affidarsi al presidente Schifani, che è commissario di tutto ma che sostanzialmente si sta caratterizzando per aggiungere ai danni della Sicilia il danno della sua inerzia personale.

Signor Presidente, ministro Locatelli, nell'ambito della Presidenza del G7, l'Italia ha promosso per la prima volta in assoluto a livello ministeriale il G7 Inclusione e disabilità, una nuova linea ministeriale che consentirà ai Paesi del G7 di confrontarsi sui temi dell'inclusione e della disabilità, di condividere strategie e impegni per contrastare le discriminazioni e garantire il diritto alla piena partecipazione civile, sociale, lavorativa ed economica. In particolare, il tema della disabilità è sempre stato affrontato nella prospettiva dell'inclusione, ma bisogna andare oltre e valorizzare la persona investendo sui talenti e sulle competenze di ognuno. In questa prospettiva è stato organizzato il G7 che potrà costituire un'occasione concreta per rafforzare gli impegni valorizzare anche l'esperienza che l'Italia sta portando avanti recentemente, adottando i decreti attuativi sulla riforma in materia di disabilità, e che molti Paesi ci riconoscono come un modello da seguire. Il G7 è stato organizzato in Umbria e si terrà il 14, 15 e 16 ottobre 2024. La prima sarà una giornata di inclusione, perché avverrà in piazza ad Assisi, con il coinvolgimento delle associazioni e delle famiglie.

Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli interroganti. Un G7 è sempre un'occasione importante e un altissimo livello di confronto tra i Paesi, ma credo che questa volta, con la linea ministeriale sull'inclusione e la disabilità, avremo un confronto ancora più importante perché parleremo di persone. volta nella storia da quando esistono questi confronti, quindi dagli anni Settanta quando sono stati creati i G7, e per la prima volta nella storia, il Governo italiano, che ha la Presidenza

possibile, per rendere davvero un'idea di condivisione, di partecipazione, di pace. Un segnale che daremo nella piazza di Assisi il 14 ottobre, dove sono invitati tutti a partecipare: anche questa è una modalità che si usa per la prima volta nella storia. Andiamo a scardinare qualche prassi, perché il 14 ottobre la stretta di mano ce la daremo come Italia insieme alle persone, insieme alle famiglie, insieme alle associazioni, insieme ai cittadini. Questo è quello che vogliamo dimostrare, ossia che l'Italia sta trainando non solo nel nostro Paese il cambiamento, con la riforma per la disabilità che mira a una prospettiva diversa, mira a valorizzare le potenzialità e non a guardare i limiti nelle persone. Diciamo stiamo scardinando davvero alcune prassi che sono consolidate anche nella presa in carico della persona con disabilità e della sua famiglia, tante complicazioni burocratiche, con la promozione ad esempio del progetto di vita e la semplificazione dell'accertamento dell'invalidità civile. Vogliamo chiederlo però anche a tutti gli altri Paesi, in Europa e nel mondo. Vogliamo fare da traino in Italia, in Europa e nel mondo per dimostrare concretezza. Non si può sempre e solo parlare, sempre e solo usare parole o filosofie per descrivere la disabilità. Noi sappiamo bene che ci sono dei problemi che riguardano anche l'integrazione sociosanitaria e la vita quotidiana, ma dobbiamo parlarne. Questo è il momento di cambiare e possiamo farlo a tutti i livelli istituzionali, anche ai più alti. Mi aspetto quindi dal G7 degli impegni concreti, che guardino anche al futuro, all'intelligenza artificiale, per esempio, oppure alla messa in sicurezza delle persone con disabilità nei momenti di emergenza umanitaria, nelle crisi delle emergenze climatiche o magari anche nei conflitti. Serve davvero una strategia condivisa su temi storici, ma anche su temi che sono attuali e molto innovativi. Il 15 ottobre ci sarà questa giornata con cinque panel, dove porteremo

Signor Presidente, ringrazio la ministra Locatelli per l'importante lavoro che sta portando avanti per far conoscere il modello italiano anche in altri Paesi e trovare accordi di collaborazione e cooperazione tra diversi Stati in modo che le persone disabili, le famiglie, i *caregiver*, ma anche gli stessi professionisti

Le famiglie e le associazioni le riconoscono il lavoro che sta facendo, come ho visto diverse volte ed anche quindici giorni fa quando siamo andati ad inaugurare Casa bella, inaugurata a Bettola, in provincia di Piacenza, per una realtà straordinaria per il Dopo di noi. sicuramente di un percorso complesso, creato grazie alla partecipazione delle associazioni, superando il mero assistenzialismo e investendo sulle competenze di ogni persona. Grazie, Ministro, per la sua risposta e per farsi ambasciatrice del modello Progetto di vita nel mondo, dando voce ad ogni persona disabile e ad ogni associazione.